in premessa evidenzio che il Ministro e i competenti uffici del Ministero, in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia, si sono attivati, fin dall'autunno del 2015, sostenendo le iniziative dei produttori vitivinicoli del Carso triestino, al fine di risolvere la problematica mediante la creazione della DOP transfrontaliera Italia-Slovenia «Teran». Rilevo, inoltre, che nell'ultima riunione del gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti del Ministero, della Regione Friuli-Venezia Giulia, delle autorità slovene e dai rappresentanti dei produttori dei due Paesi, sono stati messi a punto gli elementi tecnico-procedurali per la presentazione della domanda di protezione della DOP transfrontaliera. Peraltro, evidenzio che questo è il primo caso di DOP transfrontaliera per il nostro Paese, quindi è un procedimento nuovo e, per questo, anche particolarmente rilevante. In particolare, è stata effettuata una prima valutazione di un disciplinare comune e sono stati acquisiti elementi tecnico-storici atti a comprovare che il vitigno Terrano, registrato in Italia, è in realtà sinonimo del Refosk, registrato in Slovenia. Per uniformare il disciplinare in Italia, su richiesta della Regione Friuli-Venezia Giulia, è stato iscritto nel Registro nazionale delle varietà di vite detto sinonimo Refosk. Dopo la valutazione dei due Paesi, con il relativo esito positivo, la domanda sarà inoltrata alla Commissione europea.

In particolare, la riorganizzazione del Crea ha individuato dodici centri di ricerca, tra cui il centro di viticoltura ed enologia, cui risulta aggregato anche il gruppo di ricerca di Gorizia. Il centro cosi costituito racchiude in sé le competenze necessarie per lo sviluppo della filiera vitivinicola. La conduzione delle attività di ricerca attivate attivate presso il centro, sempre ispirata a criteri agro-ecologici e alla massimizzazione dei servizi eco-sistemici, favorisce la salvaguardia dell'ambiente e mitiga i cambiamenti climatici. Infine, il futuro laboratorio di Gorizia del centro di viticoltura ed enologia, per la sua collocazione geografica, potrà ulteriormente favorire lo sviluppo del settore vitivinicolo e raggiungere livelli di eccellenza, favorendo sinergie positive a vantaggio di tutta la filiera. replico esprimendo viva soddisfazione per la risposta e spero che il tavolo di lavoro concluda presto la sua attività. Certamente siamo anche ben felici di inaugurare una stagione di collaborazione

un'operazione e a un'attività di ricerca comune, perché è inevitabile che, essendo la vitivinicoltura al di qua e al di là di un confine che non c'è più, la collaborazione e la cooperazione

Signora Presidente, colleghi, il giorno 27 settembre 2016, come riferisce la Marina, all'atto della partenza dal porto iraniano di Bandar Abbas, la nave Euro ha condotto attività navali addestrative simboliche con la Marina iraniana. Si è trattato di attività di scambio che è consuetudine svolgere - peraltro senza interferire con le attività operative già programmate - tra le marine militari, quando si giunge o si riparte da un porto straniero ovvero durante incontri occasionali in mare. In tale contesto, le attività svolte non hanno destato sorpresa tra gli alleati. Infatti, non è stata percepita in alcun modo una flessione del tenore del rapporto bilaterale con nessuna delle marine militari dei Paesi alleati. Ciò detto, al fine di riscontrare specifica richiesta del senatore Malan, si soggiunge che non sono ad oggi previste esercitazioni militari con l'Iran. ringrazio il sottosegretario Alfano per la risposta, che ritengo rassicurante. Se davvero è una consuetudine, dobbiamo considerarla in questo modo. Soprattutto, sono rassicurato dal fatto che non sono in programma altre esercitazioni di questo genere. L'entusiasmo di alcuni esponenti del Governo per l'Iran è stato manifestato in modi assai meno usuali, e cioè con trasferte ed invito a investimenti reciproci (soprattutto italiani in Iran).

e non preludono ad altro tipo di collaborazione in ambito militare, ne sono sicuramente soddisfatto e ringrazio il sottosegretario Alfano

la difesa*. Signora Presidente, con riferimento alle problematiche ambientali relative alla laguna di Orbetello, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue. In via preliminare è opportuno precisare che le crisi anossiche e distrofiche rientrano nei processi tipici ciclici degli ambienti lagunari. La correlazione delle specifiche peculiari di questo ecosistema lagunare, con il verificarsi del raggiungimento di elevate temperature estive, ha condotto all'ingente sviluppo macroalgale avvenuto nel periodo in questione e al conseguente innesco del fenomeno distrofico. Come è noto, la laguna di Orbetello-Lago di Burano è interessata dalla presenza di quattro siti Natura 2000, la cui gestione è delegata alla Regione Toscana. Vi sono, inoltre, due riserve naturali, delle quali una statale e una regionale ed è presente, altresì, una zona umida Ramsar. Si segnala, inoltre, che, con decreto del Ministro dell'ambiente del 22 dicembre 2016, (SIC) «Laguna di Orbetello», «Duna del Lago di Burano» e «Lago di Burano» sono stati ufficialmente designati come Zone speciali di conservazione (ZSC) e pertanto su tali siti sono in vigore le misure di conservazione elaborate ai sensi della direttiva Habitat. La Regione Toscana, competente in tale ambito, ha fatto presente di aver dichiarato lo stato di emergenza regionale per l'evento eccezionale che ha interessato la laguna nel mese di luglio 2015. In fase di emergenza, come previsto dall'accordo stipulato tra la Regione stessa, la Provincia di Grosseto e il Comune di Orbetello, è stato convocato un apposito comitato tecnico-scientifico per il superamento dell'emergenza. La Regione ha evidenziato di aver provveduto al trasferimento al Comune di Orbetello delle risorse richieste per far sì che quest'ultimo potesse intervenire per la questione posta. (ARPAT), su richiesta della Regione, al fine di prevenire eventuali effetti negativi sulla qualità delle acque di balneazione ha eseguito, sempre nel mese di luglio 2015, un monitoraggio giornaliero sulle caratteristiche microbiotiche delle acque in uscita dalla laguna ed ha emesso un bollettino giornaliero con i risultati delle predette indagini. La stessa Regione Toscana ha segnalato altresì che sta elaborando una strategia sulle misure di salvaguardia e tutela della conservazione ambientale della laguna di Orbetello e questo, in particolare, con misure che recuperano e sistematizzano la disciplina già dettata per singole parti della laguna stessa, oltre a definire una disciplina di tutela per l'intero Sito Con riferimento all'area denominata di Patanella, si segnala che la stessa è stata inserita all'interno della perimetrazione del Sito di interesse con l'ultimo ampliamento avvenuto con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3.841 del 2010. Tale area è stata sede, nel corso del periodo commissariale, di un impianto di smaltimento delle masse algali rimosse dalla laguna nel periodo estivo. Nell'ambito della Conferenza di servizi del novembre 2013 è stato approvato, con prescrizioni, il piano di caratterizzazione della predetta area di Patanella. Per quanto riguarda le aree pubbliche prospicienti l'ex stabilimento Sitoco, nelle quali è stata riscontrata la presenza di silice e ceneri di piriti con metalli pesanti, sono state già valutate ipotesi di rimozione e smaltimento di tali rifiuti. Tuttavia, considerato l'enorme quantitativo da rimuovere e la difficoltà di conferimento in discarica, si stanno valutando ipotesi alternative, al fine di giungere ad una soluzione valida dal punto di vista ambientale ma anche economicamente sostenibile, in considerazione soprattutto del fatto che trattasi di aree SIC e ZPS. Questi ed altri interventi nelle aree di competenza pubblica, ad oggi interne alla perimetrazione del SIN di Orbetello-Area ex Sitoco, sono oggetto del nuovo Accordo di programma in fase di perfezionamento. Per completezza di informazione, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente ha predisposto il Piano di interventi per la tutela del territorio e delle acque, già approvato nel 2016 dalla Cabina di regia istituita il 25 febbraio 2016, e dal CIPE, nell'ambito del quale sono stati individuati, tra gli altri, anche interventi strategici e prioritari di bonifica nel SIN in questione, per un importo complessivo di circa 38 milioni di euro. In riferimento alle attività della gestione commissariale per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, si segnalano, in particolare, gli interventi di raccolta, trasporto e valorizzazione delle biomasse algali e gestione dei sistemi di riciclo idraulico.

euro per il periodo da agosto ad ottobre 2011; poco più di 289.000 per il periodo da marzo a maggio 2012; poco più di 652.000 euro per il periodo da maggio a giugno 2012;

Si segnalano altresì: i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità di accesso all'impianto di stoccaggio delle biomasse algali in località Patanella (per i quali sono stati liquidati 101.860 euro, che si aggiungono a quelli precedenti), interventi di adeguamento ambientale per l'impianto provvisorio in località Pantanella (per i quali sono stati liquidati ancora 507.127 euro), nonché i lavori di marginamento di sicurezza tra la laguna e le aree concernenti la proprietà pubblica antistante l'ex stabilimento Sitoco, ove per tale attività sono stati liquidati 134.920 euro. La gestione commissariale ha peraltro svolto attività relative alla bonifica del SIN a seguito dell'Accordo di programma stipulato tra il Ministero dell'ambiente, la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Orbetello, l'Icram ed il commissario delegato. Tali attività sono costituite sostanzialmente dagli studi e dalle progettazioni previste in apposite convenzioni. Si fa presente che il periodo commissariale è cessato con l'ordinanza di Protezione civile n. 31 il 13 dicembre 2012, per favorire il regolare subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definitivo risanamento ambientale della laguna di Orbetello. Per quanto concerne le attività del centro Ecolab di Orbetello, secondo quanto riferito dalla Regione competente, la Regione Toscana, il laboratorio è stato finanziato con i fondi pubblici della programmazione negoziata del Patto territoriale Beneficiari del contributo ministeriale sono stati l'allora commissario per il risanamento della laguna di Orbetello ed il polo universitario di Grosseto. Il laboratorio era stato realizzato per supportare le attività economiche che operano nella laguna ed anche per la gestione ambientale di un'area umida così complessa come quella in questione. Durante il periodo in cui il polo universitario è stato operativo, sono stati realizzati 42 progetti di ricerca e di attività analitiche. Con la crisi del polo universitario Siena-Grosseto, sono tuttavia venute meno per il centro Ecolab le condizioni per continuare ad operare. Con riferimento, infine, all'impianto di depurazione di Terrarossa, sulla base degli elementi forniti dal Comune di Orbetello, si evidenzia che tale impianto ha una capacità complessiva pari a 60.000 abitante equivalente. Attualmente, le quantità di reflui e rifiuti liquidi che riceve, espressi dai produttori ittici come dati di volume, superano ampiamente, dal punto di vista idraulico, le capacità dell'impianto. Tuttavia, il gestore dell'impianto ha precisato che il sistema integrato di collettamento e depurazione in questione è dimensionato per la gestione delle acque provenienti dalle itticolture

Ad ogni modo, tenendo conto degli equilibri di finanza pubblica, il Ministero dell'ambiente, unitamente al Ministero delle politiche agricole, si rende disponibile a supportare ogni ulteriore iniziativa utile alla risoluzione delle problematiche in argomento.

che gli uffici del Ministero dell'ambiente hanno fornito. Devo ammettere che è alquanto singolare e anche imbarazzante ricevere risposta a un'interrogazione con due anni di ritardo visto che chiedevamo l'intervento d'urgenza:

di tonnellate di pesci e milioni di euro buttati soprattutto in una zona dove la laguna non è soltanto turismo ma un pezzo importante dell'economia.

sono ancora necessari altri mesi evidentemente per valutare ipotesi. Capisco i costi eccessivi; capisco anche che in questo imbarazzante rimbalzo di responsabilità tra la Regione Toscana e il Comune di Orbetello sia entrato in questo momento anche il Governo,

anche attraverso il coinvolgimento di soggetti in maniera continuativa, ovvero superando le fasi commissariali che si sono succedute. Orbetello è stato straziato politicamente in tutti questi anni; addirittura abbiamo avuto per cinque anni il Ministro-sindaco, e quei cinque anni non hanno contribuito affatto a risolvere il problema drammatico della laguna. Concludo dicendo che la laguna di Orbetello è un pezzo importante dell'economia di quel territorio, territorio, che viene devastato troppo spesso anche da alluvioni e quindi ha bisogno di manutenzione, di tutela, di cura, di risorse ma anche di investimenti politici e di progetti a lungo termine. Bisogna intervenire e pensare al futuro di quella zona.

Signora Presidente, onorevoli senatori, con riferimento all'interrogazione relativa al proliferare incontrollato di alcune specie faunistiche, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente, come già evidenziato in altre occasioni, si rappresenta quanto segue. Occorre fin da subito evidenziare che sono ben noti al Ministero dell'ambiente i danni, di varia natura, arrecati in particolare alle produzioni agricole, sia in ambiti protetti così come nei territori liberi alla caccia, in particolare per quel che riguarda l'eccessivo numero di cinghiali presenti in gran parte del territorio nazionale (si stimano al momento circa un milione di individui). Al fine di poter gestire in maniera ottimale questa specie e limitarne i relativi danni, il Ministero ha ritenuto opportuno aggiornare le linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette. L'aggiornamento è stato operato in collaborazione con gli enti gestori dei Parchi nazionali e regionali. Tali linee guida rappresentano al momento il riferimento per la gestione della specie all'interno degli ambienti protetti, ponendosi come supporto agli strumenti di programmazione e regolamentazione di cui gli stessi gestori si devono dotare. Per quel che attiene il controllo numerico di fauna selvatica in esubero o problematica nelle aree protette, la legge n. 394 del lontano 1991 prevede che il regolamento del Parco stabilisca le eventuali deroghe ai divieti, prevedendo eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dallo stesso Ente parco. I prelievi e gli abbattimenti dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'ente o all'uopo espressamente autorizzato dallo stesso. Giova inoltre ricordare che, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'attività venatoria e il controllo numerico di animali selvatici in esubero o che si rendessero responsabili di danni cagionati all'ambiente sono attività distinte e non assimilabili per quanto riguarda le motivazioni, le specie oggetto di controllo, il personale impiegato e autorizzato a effettuare i controlli, nonché i metodi e i periodi stabiliti per la loro realizzazione. La stessa legge, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, prevede che le Regioni possano provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone in cui vige il divieto di caccia per svariati motivi, tra cui la tutela della produzione zoo-agroforestale, e impone che tale controllo venga esercitato selettivamente e, in prima analisi, mediante il ricorso a metodi ecologici, previo parere dell'Istituto Qualora l'Istituto verifichi l'inefficienza dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento sia in ambiti protetti di competenza regionale, che all'interno del territorio fruibile alla caccia. Pertanto, in presenza di gravi danni accertati alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica in ambienti protetti e territori liberi alla caccia, risulta coerente con la normativa vigente attuare interventi di controllo che prevedono la limitazione numerica di ungulati responsabili dei danni.

che prevedono il divieto di immissione e foraggiamento artificiale di cinghiali in natura, nonché il divieto di allevamento degli stessi in alcuni ambiti contigui a quelli protetti, con un regime sanzionatorio di natura penale per i trasgressori. Con la stessa legge è stato inoltre previsto che le Regioni e le Province autonome adeguino i piani faunistico-venatori, provvedendo all'individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale. Alla luce delle informazioni esposte, si ritiene pertanto che l'attuale quadro normativo fornisca gli strumenti idonei affinché le Regioni e le aree protette intervengano efficacemente. Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina.

un intero settore. Nel frattempo, proprio ieri, ho sottoscritto un disegno di legge a prima firma della senatrice Fasiolo (forse ne è già al corrente) sulla richiesta di nuove norme in materia di caccia al cinghiale cinghiale che evidenziano come tale problema sia diventato enorme, con danni nell'ultimo anno che arrivano anche a 100 milioni di euro, non solo alle cose ma anche alle persone.